L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

il decreto‑legge che dovremmo convertire si muove nella direzione di determinare una riduzione della popolazione detenuta. In questo senso il decreto-legge utilizza l'ordinamento penitenziario dilatando le possibilità di ammissione ai benefici e innalzando i tetti previsti dall'articolo 47-*ter* della legge la detenzione domiciliare, e sostanzialmente ampliando la possibilità di godere di misure le quali, per l'appunto, determinino una defervescenza con riferimento alla quantità della popolazione detenuta. Orbene, è chiaro (il relatore si permette di premettere questa sua considerazione alla relazione, che sarà peraltro breve) che il problema dell'eccesso della popolazione detenuta è estremamente complesso: esso trae origine dall'arsenale sanzionatorio (di questo si è discusso reiteratamente in Commissione) che è prevalentemente sbilanciato sulle pene detentive perché è l'arsenale sanzionatorio del codice Rocco, da una certa rigidità delle pene detentive conseguenti alla "riforma della riforma" (se mi è consentita questa ripetizione)

che avrebbe dovuto aprire la strada alla trasformazione degli illeciti penali minori in illeciti amministrativi punitivi (legge che, per l'appunto, non ha avuto una sua concreta attuazione), dai fallimenti reiterati delle iniziative in materia di depenalizzazione e, per toccare il tasto di maggiore rilevanza, da un eccesso di previsioni di norme penali incriminatrici. È chiaro che più il sistema si sbilancia nella direzione di prevedere fatti illeciti qualificati nelle forme del reato e puniti con pena detentiva più il problema dell'affollamento carcerario è destinato a non risolversi.

che, ad onore del vero, ancorché condivisa dalla Commissione giustizia non incide sulla materia del sovraffollamento carcerario perché è una disposizione la quale fa obbligo al giudice, allorquando dispone il provvedimento di ammissione agli arresti domiciliari, di tenere in considerazione, ma in maniera prevalente, le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Sostanzialmente, si vuole evitare che le modalità di esecuzione della custodia cautelare agli arresti domiciliari possano confliggere con le esigenze di tutela della persona offesa. Poi vi è, sempre all'articolo

allorquando verifichi che - calcolata la liberazione anticipata, calcolate le detrazioni per effetto di una precedente custodia cautelare in carcere e le eventuali, ulteriori detrazioni nascenti da dichiarazioni di fungibilità

di sorveglianza per l'applicazione della cosiddetta liberazione anticipata. L'articolo 4-*quater* poi prevede che l'emissione dell'ordine di carcerazione sarà successiva, per l'appunto, alle valutazioni in

del condannato), ma trasmetta senza ritardo al magistrato di sorveglianza le sue valutazioni e comunque il fascicolo contenente l'ordine di esecuzione. Per proseguire nella direzione segnata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, vi è poi una modifica del comma 5 dell'articolo 656

di una certa importanza (per lo meno è quello maggiormente rilevante registrato nel corso delle discussioni svolte in Commissione), Commissione), scaturito dal comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, non soltanto con riferimento ai delitti per i quali non è prevista la particolare procedura di cui al comma 5, ma anche e soprattutto con riferimento alle esclusioni della lettera *c)* del comma 9, che riguardano i recidivi, di cui al quarto comma dell'articolo 99 del codice penale. Onorevoli senatori, faccio questo discorso una volta per tutte, e dico una volta per tutte perché esso evidentemente riguarda tutta una serie di disposizioni per le quali il decreto‑legge elimina le limitazioni nei confronti dei recidivi, reiterati o specifici, alcune delle quali sono state invece reintrodotte in occasione della discussione in Commissione.

cioè, evitare che i recidivi, reiterati o specifici siano esclusi da una serie di benefici. La Commissione, ciononostante, pur consapevole non soltanto dell'importanza del problema con riferimento alla riduzione della popolazione detenuta,

che, a prescindere dai discorsi di ordine generale che sul tema della recidiva possono essere fatti - ma certamente in altra sede -, sarebbe contraddittorio collegare alla recidiva la gravità degli effetti sanzionatori preveduti dal codice penale e poi non tenerne conto in fase di esecuzione della condanna, soprattutto con riferimento a benefici che potrebbero riguardare recidivi per gravi reati, che, in relazione alla formulazione originaria contenuta nel decreto-legge del Governo e con riferimento a misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare, sostanzialmente priverebbero di significato una circostanza aggravante alla quale, al contrario, il codice penale riconosce una notevole rilevanza. In una parola, è sembrato per l'appunto contraddittorio non tenere conto della recidiva in fase di esecuzione di condanna e, ripeto, con riferimento ai benefici

dal catalogo dei delitti che non consentono il beneficio di cui al comma 5 dell'articolo 656 della fattispecie di incendio boschivo, di furto pluriaggravato e di furto in abitazione. Infatti il testo del Governo (e, a questo punto, do conto non soltanto del testo del Governo, ma anche della discussione in Commissione e di alcuni degli emendamenti introdotti) eliminava tali fattispecie dal catalogo dei reati cosiddetti ostativi

meglio noti come *stalking*, se aggravati), le due fattispecie rispetto alle quali, al contrario, si determinava l'esclusione dal beneficio.

di sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione nei confronti dei detenuti agli arresti ai domiciliari. Questo sostanzialmente è il contenuto del comma 1 dell'articolo 1, che quindi ha ad oggetto prevalente l'articolo 656 del

le modalità di esecuzione della condanna mediante il ricorso al lavoro esterno, con riferimento alla possibilità di svolgere queste attività non soltanto presso lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, ma anche presso organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. C'è poi ovviamente il legge 28 agosto 2000, n. 274, in materia di competenza penale del giudice di pace. Segue poi la lettera *b*), che concerne l'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario e la norma che concerne

(ai quali facevo precedentemente riferimento, ma in maniera riassuntiva, tant'è che adesso non ne parlerò più), perché nel decreto-legge vengono soppressi il comma 1.1, in materia di limitazione dell'entità della condanna per quanto riguarda la detenzione domiciliare per i recidivi,

un rischio di pregiudizio per la salute o le condizioni di libertà del condannato, vi sia la possibilità di chiedere di anticipare la richiesta di detenzione domiciliare proponendola al magistrato di sorveglianza anziché al tribunale di sorveglianza. poi la soppressione del comma 9 dell'articolo 47-*ter* ed il molto dibattuto riferimento

possono essere concesse solo una volta a vantaggio dei recidivi aggravati o reiterati, ovvero delle persone condannate per taluni, gravi delitti. Insomma, il numero 4)

la possibilità di consentire l'esecuzione della condanna penale (per «altri reati» si intende reati diversi rispetto a quelli connessi con lo stato di tossicodipendenza, ovvero di soggetti assuntori di sostanze stupefacenti). Pertanto, i benefici di cui al comma

ma anche agli «altri reati»: si tratta di un'espressione che alla Commissione (che ha votato un emendamento con il quale è stato soppresso l'articolo 5-*ter*) è sembrata priva di giustificazione, proprio per la ragione che essa consente un beneficio a tossicodipendenti e assuntori di sostanze stupefacenti con riferimento a reati che non trovano una giustificazione nella loro condizione soggettiva. «altri reati» è, per l'appunto, sembrata alla Commissione talmente ampia e dilatata da consentire il beneficio di cui al comma 5-*bis* soltanto in virtù di una qualificazione soggettiva e in assenza di ogni collegamento tra l'altro reato e la condizione condizione soggettiva, che, al contrario, se connessa al reato, giustifica, secondo la lettera stessa dell'articolo 5-*bis*, il beneficio della esecuzione della condanna lì prevista. Segue l'articolo 4, recante una disciplina molto dettagliata, sulla quale sono intervenuti emendamenti che poi verranno illustrati, in materia di compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo

(in particolare l'articolo 4-*bis*), volte a garantire l'efficienza dell'amministrazione penitenziaria e, in particolare, a sottrarre il numero di dipendenti dell'amministrazione penitenziaria alla riduzione della quantità del personale dipendente prevista da alcune recenti disposizioni legislative, proprio al fine di garantire, sia pure con disposizione complementare connessa, l'efficienza del sistema penitenziario. sistema deve garantire la defervescenza, la riduzione e, comunque, la qualità del trattamento, inevitabilmente non può essere vittima della falcidia della riduzione del personale dipendente disposta da alcune recenti disposizioni

Presidente, mi attengo a quanto espresso da due pronunce della Giunta e, quindi, intervengo anticipatamente in modo da consentire

ci sono degli elementi che parlano dell'esternalizzazione del lavoro e alcuni passaggi relativi all'utilizzo di queste persone per svolgere attività lavorative all'esterno del carcere con varie modalità. Io mi richiamerei qui all'articolo 98 del Regolamento richiedendo che, proprio per questa specifica particolarità, vi sia l'espressione del parere del CNEL.

e capire se questi affidati debbano avere un compenso e se svolgano un certo tipo di lavoro sociale. L'impatto c'è, e quindi io richiedo che sia allegato a questo provvedimento il parere del CNEL. *(Applausi

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, abbiamo ritenuto, come Gruppo Lega Nord-Autonomie, di presentare la questione pregiudiziale che evidenzia i profili di illegittimità costituzionale che il provvedimento reca, nonché alcune illegittimità, che vorremmo evidenziare nel merito, e tutto questo per esprimere la nostra assoluta e ferma contrarietà

quasi a regime, per affrontare il tema del sovraffollamento carcerario: in realtà, è una sorta di indulto vero e proprio, seppur mascherato. Questo provvedimento deve leggersi in linea con il successivo che arriverà, e che è stato esaminato alla Camera, il cosiddetto svuota-carceri.

cioè con atti di normazione primaria che, in teoria, dovrebbero rivestire i caratteri di straordinaria necessità e urgenza. Si tratta invece di problemi ormai cronicizzati, che andrebbero risolti con una seria politica di edilizia carceraria, con misure strutturali che il Governo deve avere finalmente il coraggio di assumere che si è tentato di assumere innumerevoli volte e che mai sono state portate a termine. In particolare, entrando proprio nel merito del provvedimento, con questo atto il Governo adotta modifiche che vanno a incidere, come dicevo, nel codice di procedura penale addirittura prorogando le funzioni e i poteri del commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, che era già previsto, integrando anche le sue funzioni e i suoi compiti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Noi chiediamo veramente dove sia il rispetto dei presupposti costituzionali di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione, che tante volte in altri provvedimenti, qui, in queste Aule, tutti richiamano. Qui il carattere di straordinaria necessità ed urgenza non ricorre. il provvedimento interviene ad inserire misure così particolari per contrastare, appunto, il sovraffollamento carcerario, andando ad incidere sull'esecuzione della pena esautorando le prerogative del Parlamento, perché si tratta di un atto di imperio assunto dal Governo. Inoltre, nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, si dice che dall'applicazione di queste misure non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato. Ma anche questo aspetto non è assolutamente chiarito, perché si pensa ad una sorta di recupero di risorse per il bilancio dello Stato, mentre in realtà dovremmo anche pensare a che cosa comporta per le finanze statali garantire la giusta e doverosa salvaguardia degli interessi dei cittadini nel momento in cui si devono comunque apprestare misure di sicurezza e protezione per coloro che sono chiamati poi a scontare

perché l'applicazione di queste norme, anche se - lo possiamo comprendere tutti - giustificata da un punto di vista sociale e morale dalla motivazione di garantire ai detenuti di poter scontare la pena in ambienti idonei,

cittadini che sono soggetti a misure personali restrittive e quanti, invece, possono usufruire del regime agevolato. Non si capisce perché alcune categorie di detenuti possano beneficiare di tali norme ed altri no. Ripeto: ciò contrasta con l'articolo 3 della Costituzione in maniera palese.

perché si interviene con un atto di urgenza (quindi con uno strumento che è quello della decretazione d'urgenza) ad assicurare al Commissario straordinario poteri ulteriori e funzioni aggiuntive, in questo caso anche esorbitando dai poteri di delega che sarebbero consentiti.

Il presente decreto-legge, poi, è anche incostituzionale, perché viola un altro principio cardine: quello sancito dall'articolo 101, primo periodo, della Costituzione, laddove recita: «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Se vogliamo infatti analizzare bene il merito del provvedimento, l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'Esecutivo in sostanza snatura la funzione legislativa del Parlamento, ossia dell'unico organo chiamato ad esercitare il volere

e non condivide neanche la questione in qualche misura sospensiva di attendere un parere del CNEL, sollevata dal collega Volpi.

i dati del sovraffollamento per intervenire, in realtà, sulla custodia cautelare. Tutto questo è vero, ma non è tutto il vero. Colleghi della Lega, con molti di voi ci siamo trovati su questi bianchi quando si è discusso dei dati del sovraffollamento. Quelli del sovraffollamento, sia quando era ministro l'onorevole Cancellieri, sia quando era ministro il collega Nitto Palma, sia quando era ministro l'onorevole Alfano sono in gran parte dati di un eccesso, di un uso e più volte di un abuso di ricorso alla custodia cautelare. mi sembra un tendenzioso ping pong - se posso permettermi di riassumerlo così - rispetto all'ancor più scivoloso ping pong nel quale si inoltra l'argomento successivo: necessità ed urgenza non ci sono perché il problema è strutturale, si tratta di un problema cronico. Credo di non essere tendenzioso come sintetizzatore o verbalizzatore del pensiero della collega. Ma questo è in qualche misura inaccettabile. È improprio di una democrazia. Finché il Senato sarà un'Aula di libertà, ciò che è necessario ed urgente per qualcuno ha eguale diritto di essere rifiutato e di essere ritenuto non necessario e non urgente da altri, per esempio dall'opposizione. E allora, smettiamola con questa droga del positivismo giuridico nel ritenere la questione costituzionale una questione kelseniana di diritto oggettivo: no, è una questione politica. E io rispetto fin da ora tutti gli argomenti di merito, di opposizione, se del caso di ostruzionismo, ma non accettiamo come Gruppo di antica tradizione democratica che la questione costituzionale subentri furbescamente alle questioni del merito politico. Un'ultima considerazione che vale, in qualche modo, ad assorbire nella questione pregiudiziale gli argomenti a base della richiesta del parere del CNEL, questione in qualche misura sospensiva, avanzata dal senatore Volpi. Ma se questo provvedimento tocca un meccanismo basato sui lavori socialmente utili, forse un meccanismo di costi, da questo punto di vista l'articolo 81 della Costituzione applicato alla conversione di un decreto-legge ha tutt'altre modalità Senatore Volpi, la funzione della pena nella nostra Carta costituzionale non è una funzione meramente afflittiva e, quindi, l'argomento dei lavori socialmente utili si innesta a buon diritto. Pertanto, da questo punto di vista, ripeto quello che ho detto in ordine agli argomenti sollevati ci sono occasioni di merito nelle quali farlo valere. Non nascondiamoci dietro una questione costituzionale che non c'è e manteniamo tutto il diritto, in sede politica, di legiferare su questa materia. Lo stesso vale per quella che mi è sembrata - me lo consenta la collega - la consueta e abusata furbizia della Costituzione sull'eguaglianza. Arrivare con un'abile torsione degli argomenti a regalare una condizione di privilegiati, in positivo rispetto all'ordinamento, a chi è in carcere mi sembra una argomentazione troppo intelligente per non sembrare troppo furba e, quindi, estranea al dettato, allo spirito e alle norme della nostra Costituzione.

sollevata dalla Lega, condividendone sostanzialmente le osservazioni di fondo, ovvero la censura dell'ennesimo ricorso alla decretazione d'urgenza, in deroga alla lettera e allo spirito dell'articolo 77 della Costituzione, che costringe ancora una volta (e temiamo che non sarà l'ultima) questo Parlamento e anche le Commissioni a dover rincorrere l'esame e un'analisi, che per questi motivi molto spesso non può essere neanche approfondita e ben ponderata, di tutto l'articolato normativo. Ancora una volta ci troviamo a dover fronteggiare provvedimenti normativi, per quanto ipoteticamente necessari - e la questione carceraria, lo sappiamo benissimo, esiste e merita una soluzione dignitosa per un Paese che vuole ancora considerarsi civile -

la questione pregiudiziale QP1 non è stata formulata come una questione di costituzionalità, anche se uno dei primi argomenti è quello della violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Ricordo a me stesso che lo scrutinio di costituzionalità di una norma si fa rispetto ad un'altra norma e non rispetto a modifiche legislative della situazione pregressa; altrimenti tutto sarebbe incostituzionale, perché avremmo un paragone tra la nuova e la vecchia disciplina e non tra due norme esistenti. Non si può poi ragionare in termini probabilistici rispetto ad un disegno di legge di conversione di un decreto-legge che fissa alcuni paletti dal punto di vista

un'attività ben specifica e disciplinata. Il provvedimento in esame serve a garantire una più spedita funzionalità e a realizzare un minimo di dignità nelle carceri.

La critica al decreto-legge, e quindi al ricorso alla decretazione d'urgenza, pur trovandomi d'accordo in generale, nell'ipotesi specifica non regge.

un ulteriore corollario del sistema complessivo di gestione dei penitenziari e delle carceri, che dunque va considerato unitariamente. Per quanto concerne la questione chiamiamo sospensiva, di parere del CNEL «quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale». Pretendere che il lavoro volontario e gratuito dei detenuti, ove possibile, che rappresenta un'esplicitazione concreta del dettato costituzionale, possa incidere sulla

Si tratta però di un lavoro volontario, gratuito, che serve alla risocializzazione e alla rieducazione del condannato, per cui non capisco quale possa essere la valutazione del CNEL. Per tali ragioni, quindi, anche

Signor Presidente, il collega Caliendo ha già ampiamente sviluppato il tema concernente gli aspetti strettamente connessi con l'attività lavorativa che potrebbe potrebbe analogicamente giustificare l'intervento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ma l'ha giustamente escluso in quanto riguarda attività lavorativa volontaria non retribuita di detenuti. Quindi è un caso a sé,

determinata dalla condizione di sovraffollamento, che ha previsto interventi straordinari sia in sede legislativa sia da parte del Presidente

In questo contesto, anche nella sentenza che sviluppa tale argomento, più nota come sentenza Torreggiani, questi temi sono strettamente connessi con l'orientamento suggerito agli Stati membri di depenalizzare, ove possibile, e quindi di introdurre elementi diversi dalla carcerazione

per sopperire al sovraffollamento è anche previsto - un Commissario straordinario è incaricato di questo ruolo

Signor Presidente, sono essenzialmente cinque i motivi a sostegno della pregiudiziale di costituzionalità che sono stati illustrati e presentati per iscritto, riguardano, in sintesi, gli articoli 77, 76, 3, 81 e 101 della nostra Carta costituzionale. Rispondendo alla prima parte delle contestazioni, quelle relative all'articolo 77, ovvero alla sussistenza o no dei requisiti di necessità ed urgenza, credo sia sufficiente richiamarsi alla tematica di cui stiamo trattando per renderci conto, invece, che ci troviamo in una vera e propria situazione di emergenza. Quando se ne parla a livello nazionale - in tutti gli ambiti: sociali, politici ed istituzionali - ci si rende conto tutti quanti del fatto che il sovraffollamento penitenziario rappresenta un'emergenza nazionale, è una questione urgente per una serie di motivi che non vengono assolutamente posti in discussione da alcuno. Proprio il decreto-legge in esame viene proposto al Parlamento dal Governo come una prima soluzione nell'ambito di una serie di soluzioni che devono essere affrontate, discusse e votate per cercare di sopperire alla situazione ed eliminare questa piaga sociale e istituzionale.

esistono sentenze e provvedimenti di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti del nostro Stato che impongono in tempi brevi, se non addirittura brevissimi, un rimedio o comunque proposte di soluzione.

che intervengono sul codice penale, su quello di procedura penale e su leggi speciali come quelle in materia di sostanze stupefacenti, per cui non ravviso una questione di delega in senso tecnico a norma dell'articolo 76. Pertanto, anche da questo punto di vista la contestazione andrebbe rigettata. Così come andrebbe rigettato il riferimento all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, perché non si ravvisa assolutamente, da parte nostra, una violazione del principio di uguaglianza sancito da questa norma costituzionale. È indicato invece espressamente un profilo di ragionevolezza, perché con questo decreto-legge si interviene su determinate situazioni effettuando una cernita molto puntuale e precisa tra coloro che sono caratterizzati dalla specifica condizione dell'allarme sociale e coloro che invece, proprio perché non dotati di questa caratteristica in quanto non presentano profili di allarme sociale, vengono, per così dire, beneficiati da questo provvedimento. Quindi, la logica intrinseca del disegno di legge è chiarissima: si interviene per determinate situazioni di

toccata. Proprio per questo il provvedimento si muove su una doppia linea di intervento: da un lato, ci sono le misure dirette a incidere strutturalmente sui flussi carcerari, che agiscono sugli ingressi sia in uscita che in entrata; dall'altro, si prospettano maggiori opportunità di trattamento alternativo al carcere per i detenuti meno pericolosi, proprio per andare incontro alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

mi risulta francamente incomprensibile, perché fa riferimento all'articolo 101, primo periodo, della nostra Carta costituzionale, in cui si dice che «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Non comprendo come questo decreto-legge

che riguardano l'intervento su persone detenute, caratterizzate da più o meno grave allarme sociale. Certamente ci sono questioni che riguardano la fase riabilitativa, di rieducazione. La disposizione, quindi, consentirebbe a queste persone di passare al lavoro e di utilizzare al meglio il loro tempo nell'ottica sociale del recupero perché, sappiamo tutti benissimo, che, dove ci sono possibilità di lavoro per i detenuti, il tasso di recidiva crolla in maniera incredibile (credo sia superiore all'80 per cento). Questo è un dato sociale, politico e anche economico estremamente importante da ricordare. Su questo punto, come ricordato, mi limito a dire che l'articolo 2 di questo decreto-legge prevede che «i detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività...(...)». Sono, quindi, esclusivamente attività in vantaggio. Non vedo come

fa riferimento ai limiti già contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2012 e si limita alla precisazione di compiti che sono finalizzati esclusivamente

Signor Presidente, innanzitutto mi permetto di rivolgere un ringraziamento al Sottosegretario presente che rappresenta il Governo, anche perché, per questo provvedimento urgente e importante, per cui bisogna fare le corse per liberare detenuti, non vedo in quest'Aula, come sta capitando per molti provvedimenti, il Ministro.

collega Sottosegretario rappresentare il Governo su due provvedimenti diversi. Chiederei ai colleghi di maggioranza di sollecitare i Ministri a venire in questa Aula.

Signor Presidente e onorevoli colleghe e colleghi, ho ascoltato con grande interesse l'intervento del collega leghista e le riflessioni che lo hanno portato a fare simili dichiarazioni. Dal punto di vista politico ognuno di noi è libero, all'interno di quest'Aula, di sostenere le proprie tesi, di cercare con forza di dimostrare che sono giuste e convincere i colleghi ad intraprendere una strada che consequenzialmente porta ad un voto e alla scrittura di una legge. Vorrei fare alcune riflessioni, e chiedo al Presidente di autorizzarmi, nel caso in cui non riuscissi a completarle, a consegnare il

Signor Presidente e onorevoli colleghe e colleghi, alcuni di voi conoscono meglio di me la storia delle carceri nella modernità. Alcune ed alcuni di voi forse avranno letto «Sorvegliare e punire» di Michel Foucault. Si tratta dello stesso pensatore europeo di origine francese che ha scritto «La nascita della clinica» e che ha tenuto le memorabili conferenze sulla cura di sé e la conoscenza di sé. Per questo filosofo vi è un sotterraneo di millenari parallelismi fra i processi di individuazione, sorveglianza, prevenzione e punizione di ogni deviazione dalla norma che i popoli-nazioni e gli Stati storicamente istituiscono, conservano e modificano. Il carcere e la clinica nella modernità sono le istituzioni di contenimento dei devianti, i luoghi per difendere le collettività e le comunità dalla violenza e dal contagio dei comportamenti di quei simboli che non sono in grado di avere cura, né conoscenza di sé. L'altro nome popolare del carcere è "galera". La galera era una nave ancorata al largo dove erano rinchiusi i segnalati, i sospettati, gli imputati in attesa di un processo e di eventuale condanna; nel qual caso il condannato veniva prelevato e condotto all'esecuzione della pena. Ma già nel Settecento la macchina di sorveglianza e punizione si inceppò, tanto che Jeremy Bentham, filosofo europeo di origine britannica, riformatore, economista e giurista insigne, e con lui ogni suo allievo sparso per le capitali d'Europa, dedicò oltre la metà della sua longeva attività di pensatore al problema della convivenza civile connessa alle sue ombre connaturate: malattia e reati, clinica e galera. Nel 1791 pubblicò addirittura un progetto di carcere ideale, osservatorio totale, una casa di ispezione continua: si trattava di una struttura le cui celle singole erano disposte a semicerchio con cancelli aperti verso il centro, in modo che la luce proveniente dalle finestre rendesse visibile ad un singolo sorvegliante posizionato al centro la vita di ogni detenuto 24 ore su 24. Era l'ossessione della sorveglianza totale e continua come punizione di per sé, la privazione di qualsiasi spazio privato: il reo e l'ammalato non avrebbero dovuto avere alcuna intimità. Fortunatamente, dalla Rivoluzione francese ad oggi abbiamo scoperto, rivendicato, istituzionalizzato e difeso i diritti umani come bene inviolabile anche dell'ammalato e del reo. Abbiamo cominciato a sperare sulla possibilità della redenzione del reo e della guarigione dell'ammalato. Accanto alla difesa della collettività, alla sicurezza, abbiamo istituzionalizzato il trattamento individuale e il reinserimento sociale. In Europa, e forse nel mondo, grazie ai nostri connazionali toscani siamo stati i primi ad abolire la pena di morte. Dall'opera «Dei delitti e delle pene» di Cesare Beccaria alla legge n. 663, del 10 ottobre del 1986, detta legge Gozzini, dal nome del senatore Mario Gozzini che ne presentò il disegno di legge, abbiamo, almeno sulla Carta costituzionale, il migliore sistema che connette sorveglianza e punizione. Sul fronte della clinica, con la legge n. 180 del 13 maggio 1980 (sulla salute e sulle malattie mentali), la legge di riforma n. 833 del 23 dicembre 1978, che istituì il Servizio sanitario nazionale, n. 229 del 1999 (riforma sanitaria-*ter*), abbiamo cercato di inserire i diritti della persona nei processi di sorveglianza e punizione. Sulla carta appunto, nella realtà abbiamo solo poche istituzioni appropriate. Lungo i quattro lustri appena trascorsi avremmo voluto fare ulteriori passi avanti verso la destatalizzazione e la responsabilizzazione delle istituzioni civili e sociali. dei responsabili), interessi privati, commerciali, partitici e politici, ignoranza e pressapochismo, principianti arroganti, persone di buona volontà ma ingenui, crollo repentino di ideologie granitiche, hanno concorso nel vanificare le liberalizzazioni e le socializzazioni, facendo fare passi indietro pseudostatalizzanti. Ci troviamo così ora con istituzioni penitenziarie al collasso e persone detenute costrette a sopravvivere in condizioni inumane, da una parte, e, dall'altra, con un sistema sanitario fra i migliori del mondo ma con lo stato di salute della popolazione al quarantesimo posto

un terzo di tutti i detenuti sono in attesa di giudizio. Circa 20.000 sono in carcere per reati di microcriminalità connessi ai comportamenti conseguenti alla malattia della tossicodipendenza. Abbiamo circa 100.000 procedimenti all'anno che cadono in prescrizione perché i magistrati non sono in grado di ottemperare in tempi utili alla obbligatorietà dell'azione penale. Secondo alcune ricerche della Confindustria le mancate giustizie ci costano quasi il 7 per quando non si riusciva a venire a capo né della sorveglianza, né della punizione, si ricorreva alla religione; secondo il filosofo e politico Crizia poiché anche gli uomini probi avrebbero commesso reati, se certi di non essere visti e di restare impuniti, allora qualcuno ebbe l'idea di creare un dio che osservasse il comportamento di ognuno anche nel segreto della propria mente D'altra parte, nella Sacra Bibbia, via via che il popolo di Dio costruisce la propria storia, si evolve il concetto di sorveglianza e punizione, di "Seddaqah": un concetto di punizione che è risarcimento sociale e reinserimento come processo per la sicurezza della comunità. Un concetto che ha in sé l'idea che solo la socializzazione potrebbe avere risorse per la trasformazione del reo in un cittadino socialmente utile. Non più la vendetta dei più sul singolo, della società sul deviante. La conversione in legge del decreto n. 78 del 1° luglio 2013 di cui stiamo discutendo, centrandosi sull'estensione (quantitativa e qualitativa) delle misure alternative alla pena e alla custodia in carcere, sia nella fase di esecuzione che di rinvio a giudizio, mi pare che tenga conto di quei momenti di civilizzazione di cui mi sono permesso di dar cenno e, particolarmente verso la socializzazione, la territorializzazione e domiciliazione del carcere; condivido ovviamente anche quei punti

come scrisse nell'omonima enciclica Giovanni Paolo II, dunque, voterò a favore della conversione in legge del decreto n. 78 del 1° luglio 2013 e pongo la mia fiducia sulla capacità di tenuta ed intelligenza del Governo nell'affrontare alcune delle cause che stanno a monte dei ricorrenti affollamenti, mettendo mano, per esempio, ad alcuni dei temi per i quali i radicali, ed altri parlamentari si sono battuti all'interno e fuori di quest'Aula insieme al PdL.

in prima battuta vorrei sottolineare che il nostro Paese per il problema delle carceri è stato richiamato anche dalla Commissione europea, e lo stesso Capo dello Stato ha voluto

come può sentirsi un servitore dello Stato quando la risposta della politica è sommaria, pressappochista e senza

coinvolgendo uno dei più grandi architetti a livello mondiale, Norman Foster, che riproponeva lo stesso volume in verticale, creando un elemento di riconoscimento all'interno della città.

Questo è successo: un funzionario dello Stato si è messo di traverso quando legittimamente un sindaco e un Ministro hanno tentato di fare a Milano un'operazione grandiosa, come si fece a suo tempo per la Fiera.

colleghi, anche in questa legislatura, puntuale come le tasse, si ripropone l'annoso problema del sovraffollamento delle carceri. Come al solito, in questo Paese non curiamo le cause, ma interveniamo soltanto sulle conseguenze dannose. Sappiamo bene che questo Paese non può permettersi di abolire il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, non è maturo, e mi rendo conto che questo Governo non potrebbe mettere mano senza scosse al sistema delle pene, perché non è sufficientemente forte. Il nostro è un sistema imperniato sulle cosiddette leggi Bossi-Fini e Fini-Giovanardi, due pessime leggi che hanno dato una pessima prova, contribuendo in modo decisivo a riempire le carceri di poveracci che chiedono solo di essere curati o di poter vivere del proprio lavoro, qui o altrove, visto che nella loro patria non possono farlo. Detto questo, non rimaneva che risolvere il problema empiricamente. Occorreva trovare un posto dignitoso per ogni detenuto. A questo avrebbe dovuto servire, per esempio, l'articolo 4 del decreto-legge oggi al nostro eppure questo provvedimento non individua soluzioni, ma potenzia una struttura, il commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, che non serve a niente. La soluzione al problema del sovraffollamento delle carceri esiste già. Un magistrato tenuto in grande considerazione, a parole, da questo Governo, Nicola Gratteri, ci ricorda che ci sono sistemi molto semplici per svuotare le carceri. Nessuno ancora ha spiegato perché nel 1994 sono state chiuse le carceri nelle isole di Pianosa e dell'Asinara. In Italia ci sono carceri militari vuote: perché queste cose non le diciamo? In molte carceri ci sono bracci vuoti: perché non ripristinarli e utilizzarli al meglio? Da questo disegno di legge, poi, mi sarei aspettato una indicazione precisa che mi chiarisse, ad esempio, il destino del carcere di Gela, inaugurato già tre volte e oggi aperto per 32 detenuti. E che ne è del carcere di Arghillà in Calabria, una struttura all'avanguardia, ora che la strada per arrivarci è stata costruita? Andrà a regime? E il carcere di Cropani? E quello di Irsina? Evito di elencarli tutti, ma da un conteggio recente risultano ancora una trentina le carceri vuote, che potrebbero essere utilizzate per risolvere il problema del sovraffollamento in breve tempo. E che dire infine del personale carcerario? Il disegno di legge si preoccupa di reperire e/o costruire alloggi per il personale, che però è insufficiente. Si pensa di adeguare gli organici? Ancora una volta nessuna risposta. Cari colleghi, non possiamo più permetterci guerre sante alla droga o allo straniero che sbarca nel nostro Paese in cerca di pane e di lavoro. Se anche aprissimo nuove carceri, non potremmo impegnare a lungo, in questi tempi di crisi, tante risorse. Questo provvedimento non rappresenta un passo in avanti ma un passo laterale. Seppur non completamente bocciabile, non risolve praticamente nulla. Consideriamolo un punto di partenza, per decidere che tipo di Paese vogliamo diventare. Potremmo costruire un Paese di cui essere orgogliosi, accogliente e misericordioso termine è inteso come sentimento di compassione e pietà per l'infelicità e la sventura altrui che induce a soccorrere, a perdonare e non a infierire); un Paese che, con buona pace dei contabili, ci costa pure meno. Prevenire funziona molto meglio che curare.

innegabilmente a incidere sulla vita dei nostri concittadini. Francamente, parlare di redenzione, come abbiamo sentito fare in questa circostanza, sa molto di ipocrisia perché si mette in relazione la redenzione del detenuto con la necessità di dare più spazio nelle carceri.

E qui ha ragione chi viene ad argomentare che, per l'ennesima volta, si provvede con l'urgenza di un decreto-legge a una situazione che è diventata insostenibile. Questo Paese, infatti, sembra abituato ad intervenire solo con i decreti e sulle urgenze, proprio per l'incapacità di guardare i problemi e risolverli anzitempo. È su questo aspetto che dobbiamo iniziare a soffermarci. Occorreva un decreto-legge? Occorreva un intervento così forte, quando invece, come è già stato bene argomentato, si possono costruire piani che diano anche spazio all'economia? Ha detto bene prima il senatore Crosio, quando ha fatto l'esempio del Comune di Milano: la stessa struttura carceraria può essere un'opportunità di investimento nel nostro Paese. Si rimodellino queste carceri, che sono obsolete e spesso ottocentesche, ma non svuotandole dei detenuti che sono al loro interno, bensì mettendo a disposizione strutture carcerarie adeguate ad un Paese che si dice civile.

quanto meno surreale. Il senatore Casson parlava di piaga sociale del sovraffollamento, ma io dico che la piaga sociale è la lentezza dei processi che lascia per anni i cittadini in attesa di giudizio all'interno delle carceri. Piaga sociale sono i delinquenti recidivi che squassano la vita dei cittadini onesti. E piaga sociale è anche un mondo politico che non riesce a dare una risposta coerente con le aspirazioni di onestà che i nostri cittadini hanno. Quale messaggio di inaffidabilità diamo poi alle forze dell'ordine?

la soluzione non è stata trovata perché, dopo neanche due anni dall'ultimo indulto, ben 20.000 detenuti sono tornati in carcere. Quindi, il problema del sovraffollamento c'è e rimane.

tipo. Perché non avete portato avanti quei progetti di edilizia carceraria che erano stati messi in piedi dall'allora ministro leghista Castelli? Si parla del problema del sovraffollamento, ma non si fa nulla per realizzare nuove carceri. Invece pensate a provvedimenti tampone come questi, che - come è stato detto anche dai miei colleghi

Lega Nord. Il provvedimento - continuiamo a ribadire e ad insistere su questo concetto - incide sulla messa in prova, in quanto introduce una misura che è dannosa perché non tiene conto della necessità che le pene siano effettivamente scontate, soprattutto per reati e crimini particolarmente pericolosi,

Quindi chiediamo che il Governo, se davvero vuol risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, si impegni ad insistere a portare avanti e proseguire politiche di accordo bilaterale con i Paesi di provenienza dei detenuti stranieri, così riuscirebbe a risolvere da subito e in maniera efficace e concreta questo annoso problema.

ci apprestiamo a convertire in legge affronta un'emergenza gravissima, che ci è costata la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione della norma che vieta la tortura e i trattamenti inumani, e lo fa, a differenza di quanto sostiene la Lega, non cedendo alla tentazione dei tagli lineari o con provvedimenti quali l'indulto e l'amnistia (che non rimuovono le cause del problema e fanno sì che questo sia

riaffermare il primato costituzionale della finalità rieducativa della pena, eliminando gli automatismi ed affidando alla valutazione discrezionale del magistrato il trattamento punitivo che deve poter essere individualizzato, incide non soltanto sulla consistenza e la dimensione della popolazione carceraria - il tema che stiamo affrontando

cento per coloro che vengono immessi nel circuito lavorativo. È un dato che fotografa la peculiarità della nostra situazione in rapporto a quella di altri Paesi europei. È un dato che i condannati ammessi alle misure alternative in Inghilterra sono 197.000, in Spagna 111.000, in Germania 120.000, in Francia 123.000, mentre in Italia sono 13.000. Noi dovremmo, semmai, fare di più. Dovremmo eliminare le preclusioni normative all'accesso alle misure alternative al carcere previste dall'articolo 4‑*bis* dell'ordinamento penitenziario, stratificatesi nel corso di reiterati interventi del legislatore indotti dall'allarme sociale provocato da alcuni reati, e ricondurre la norma alla sua *ratio* originaria di prevenzione relativa ai soli condannati per delitti di matrice mafiosa e di terrorismo, sulla base della ragionevole presunzione di rilevante pericolosità di tali soggetti, correlata al perdurare di collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento.

siano effettivamente scontate in carcere, impegna il Governo a considerare la necessità di incidere sul sovraffollamento carcerario proseguendo ed ulteriormente sviluppando la politica di sottoscrizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei detenuti stranieri, con riferimento ai paesi da cui provengono complessivamente quasi il 40 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro Paese di origine Purtroppo, prendiamo atto che, con l'insediamento di un Governo composto da una forte maggioranza di sinistra, ricompare sempre il solito problema: dobbiamo liberare i criminali. Si riducono i fondi per le forze dell'ordine che tutelano il cittadino e si rimettono in circolazione i criminali. Chiamiamolo svuota carceri, chiamiamolo indulto, chiamiamolo amnistia, ma il vostro scopo è liberare i criminali. Vi preoccupate dei diritti e della dignità dei carcerati e vi disinteressate di garantire i diritti e la dignità delle vittime dei reati commessi da questi criminali. Ho detto Governo di sinistra, ma ricordo che anche PdL e Scelta civica ne sono complici. Non ricordate forse che più del 20 per cento dei detenuti liberati con forti sconti di pena è ritornato in carcere per aver ripetuto lo stesso reato entro un anno? Ricordando che quasi il 40 per cento dei detenuti è composto da stranieri, la Lega Nord è fermamente convinta che questi debbano scontare la loro pena nel Paese di origine. Ma a voi questo interessa poco. È più facile liberare i criminali, che poi voteranno per voi, che tutelare i cittadini onesti. Diamo pure i domiciliari agli extracomunitari, che dopo due giorni saranno già scappati per commettere altri reati in giro per l'Italia. Per l'interesse dei vostri amici, state dando licenza di delinquere. Sotto quella veste da falsi buonisti state solo garantendo l'impunità per i criminali e dimostrate tutto il vostro disinteresse nei confronti dei cittadini onesti. Ogni giorno sbarcano sulle nostre coste centinaia, per non dire migliaia, di clandestini che nel giro di poco tempo saranno a vagabondare per l'Italia senza reddito e che quindi per vivere dovranno dovranno scippare e diventare spacciatori e voi avete ben pensato di permettere a queste persone di essere libere. Avete presentato questo provvedimento per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri ma, secondo voi, è questo il modo di gestire la giustizia in una Nazione?

Questi provvedimenti sono misure tampone che cercano semplicemente di ridurre con piccoli interventi un problema grosso, un problema che non va assolutamente affrontato in questa maniera. Nel decreto‑legge si parla ancora di proroga dei poteri del commissario per l'edilizia carceraria. Devono essere costruiti nuovi istituti, devono essere approntate tutte le iniziative atte a risolvere il problema delle carceri, ma questo non è il metodo. Queste sono delle soluzioni veramente all'italiana che porteranno a conseguenze all'italiana. Io però mi pongo solo e semplicemente una domanda: non non è forse ipocrita pensare di strutturare il numero dei reati in funzione delle dimensioni delle carceri e non le dimensioni delle carceri in funzione del numero dei criminali?

con un'eccedenza della popolazione carceraria di 20.000 posti nei 206 istituti penitenziari italiani, istituti troppo spesso fatiscenti e inadeguati. Ma il sovraffollamento non completa la grave situazione di emergenza: dobbiamo aggiungervi la carenza di attività trattamentali, che dovrebbero rappresentare lo strumento per dare attuazione alla funzione rieducativa della pena, come disposto dall'articolo 27 della Costituzione. La mancanza di attività trattamentali contribuisce infatti ad una espiazione della condanna in solitudine, che troppo spesso è causa degli oltre 71 suicidi l'anno. Non possiamo pertanto illuderci che siamo di fronte ad una delle tante emergenze del nostro Paese, che possa essere affrontata soltanto con provvedimenti di clemenza; si tratta piuttosto di un problema strutturale che caratterizza da 20 anni il sistema penitenziario e penale del nostro Paese. Non è sufficiente il piano carceri del 2010 e non è sufficiente la conversione del decreto-legge n. 78 al nostro esame per ripristinare una normalità che è sì giuridica ma prima di tutto umanitaria e che attiene alla salvaguardia della dignità dell'uomo, ai suoi diritti, e attiene al livello di civiltà che un Paese moderno dovrebbe garantire ai detenuti e a chi nelle carceri lavora, come il Corpo della Polizia penitenziaria. Questi ne sono però i primi passi. Prioritario è infatti l'intervento volto ad evitare il fenomeno delle porte girevoli, ovvero dei troppi ingressi in carcere per brevi periodi, così come l'eccessivo ricorso alla custodia cautelare: cento dei detenuti è infatti in attesa di giudizio definitivo, e di questi il 17 per cento verrà assolto ed avrà diritto al risarcimento per ingiusta detenzione. Allora, appaiono dovuti i richiami e le condanne dell'Italia da parte della Corte europea di Strasburgo per violazione dei diritti umani: oltre 14.000 denunce e 200 condanne. La riforma del sistema di giustizia è urgente: riforma per una giustizia indipendente, efficiente, che possa creare quel clima di fiducia e di stabilità che è anche il presupposto per attrarre investimenti produttivi. Manifestiamo pertanto il nostro apprezzamento per questo primo intervento di legge che modifica il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario, al fine di rafforzare l'ammissibilità e l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ed eliminare ostacoli giuridici ed automatismi di divieti

come ci mostrano le statistiche dei recidivi detenuti; la liberazione anticipata già in fase di ordine di esecuzione; l'innalzamento a quattro anni del limite per l'ammissibilità alla detenzione domiciliare; l'estensione dell'articolo 21 della legge 26 luglio per il lavoro all'esterno retribuito anche ai casi di lavoro di pubblica utilità e di volontariato; l'abrogazione dei divieti automatici; i maggiori poteri al magistrato di sorveglianza per l'applicazione provvisoria dei benefici stessi. Dovranno essere liberati 20.000 posti per stessi. Dovranno essere liberati 20.000 posti per disposto della sentenza Torreggiani della Corte di Strasburgo entro la primavera del 2014. L'orizzonte su cui lavorare in futuro, per superare un sistema attuale dell'esecuzione penale che ci appare meramente punitivo e vagamente rieducativo, dovrà essere quello di virare verso una giustizia che che contribuisca allo sviluppo di una coscienza di responsabilità del reo, riparativa nei confronti della vittima, ma soprattutto nei confronti della collettività; un sistema che estenda la messa alla prova sia in fase processuale che in esecuzione penale e che consenta l'individualizzazione del trattamento anche con forme di custodia attenuata in circuiti penitenziari differenziati; un sistema dove il carcere sia sempre meno preventivo e dove i tempi di trattazione e di indagine siano garanzia del giusto processo. Queste sono le tappe che ci attendono ancora.

sovraffollamento carcerario e all'inadeguatezza delle strutture penitenziarie. Parliamo dell'inadeguatezza di chi dovrebbe fare scelte in ordine alla sicurezza del Paese e dare tempi certi all'azione della giustizia, lenta nel sentenziare e che riempie le carceri di detenuti in attesa di giudizio.

che affrontano i viaggi della speranza, richiamati da quella parte politica oggi assente in Aula (come si può osservare) che usa temi di bandiera per un proprio tornaconto. la falsa illusione di un lavoro che non riescono più ad avere nemmeno i nostri figli e le nostre famiglie. Avete preso coscienza della reale situazione economica e sociale del nostro Paese? pene più severe, certezza nella loro applicazione, il coraggio di affrontare il problema dell'immigrazione irregolare confermando l'aggravante legata alla condizione di clandestinità, per contrastare concretamente il nascere di sacche sociali di emarginati, ai quali come unica possibilità resta quella di delinquere.

riempirete ancora i centri di assistenza fino allo sfociare di inevitabili episodi di criminalità? È inutile svuotare carceri che in poco tempo saranno nuovamente sovraffollate, portando ad una situazione esplosiva di contrasti sociali.

Interventi concreti in materia di sicurezza avevano fermato il fenomeno dell'immigrazione clandestina colpendo anche chi ha utilizzato questi immigrati per il proprio tornaconto, datori di lavoro che li hanno sfruttati ed emarginati. Scontare la pena nel Paese d'origine, la procedura di espulsione e il rimpatrio immediato sono una tutela e una sicurezza per le famiglie che vivono nella legalità, rispettano le regole e hanno il diritto quindi di essere rispettate dalle istituzioni. Signori del Governo, abbiate il coraggio di stipulare gli accordi con gli Stati esteri per far scontare le pene agli stranieri nei loro Paesi d'origine. Abbiate il coraggio di scelte audaci per la tutela dei vostri cittadini.

sull'esecuzione della pena per portare all'attenzione dell'Aula e del Governo anche la gravissima situazione penitenziaria della Liguria, come esempio per tutta Italia. Le cifre del sovraffollamento ligure (al 30 aprile 2013) sono drammatiche: in Liguria ci sono 1.889 detenuti, di cui 72 donne e 1.817 uomini; 781 sono in attesa di un giudizio definitivo e 1.107 sono condannati.

In Liguria resta altissima la presenza di detenuti stranieri (tra il 55 e il 65 per cento dei presenti a seconda degli istituti) e dei tossicodipendenti (oltre il 30 per cento dei presenti, rispetto ad una media nazionale che si mentre sono solamente il 17 per cento i detenuti che lavorano, peraltro in servizi di istituto, e per di più per poche ore al giorno. I detenuti non sono impiegati in attività lavorative o utili alla società (come i lavori di pubblica utilità) e restano chiusi in cella in media venti ore al giorno, alternandosi tra chi sta seduto e in piedi per mancanza di spazio; questo favorisce l'ozio in carcere e l'acuirsi della tensione, che si tramuta in risse, aggressioni, suicidi e tentativi di suicido, rivolte ed evasioni. A sua volta, questo genera condizioni di lavoro dure, difficili e stressanti per la Polizia penitenziaria, che sappiamo essere sotto organico. Nell'anno 2012, nelle sovraffollate carceri liguri, i detenuti si sono resi protagonisti di 92 atti di autolesionismo (e cioè ingestione di corpi estranei come chiodi, pile, lamette; tagli diffusi sul corpo e provocati da lamette) e 29 tentativi di suicidio. Sono state 93 le colluttazioni e 19 i ferimenti. Sono state 5 le evasioni in Liguria da parte di altrettanti detenuti che non sono rientrati in carcere dopo aver fruito di permessi premio e semilibertà. Nel corso dell'anno, infine, sono stati complessivamente 6.000 i detenuti della Liguria che hanno dato luogo e partecipato alle molte manifestazioni di protesta collettive sulla situazione di sovraffollamento delle carceri e sulle critiche condizioni intramurarie. Perché i detenuti possano lavorare, occorre una legge apposita e la volontà politica per farla. Le statistiche ci dicono che il condannato che espia la pena in carcere ha un tasso di recidiva del 68,4 per cento contro il 19 per cento di chi ha fruito di misure alternative e addirittura l'1 Altro dato significativo della Liguria riguarda il «carcere invisibile», ossia le misure alternative e di sicurezza e le altre misure sostitutive della detenzione, che coinvolge complessivamente in Liguria oltre mille persone. Oggi abbiamo in Liguria 448 persone affidate in prova ai servizi sociali: di queste, circa 150 sono tossicodipendenti, 28 fruiscono di semilibertà, 239 di detenzione domiciliare, 115 di libertà vigilata e 214 di altre misure, tra le quali quella del lavoro di pubblica utilità per i soggetti (209) sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. Conoscendo questa situazione gravissima che riguarda la Liguria, ma che evidentemente interessa tutto il nostro Paese, ho presentato l'ordine del giorno G101, le cui proposte hanno carattere assolutamente nazionale. È evidente che scontare la pena fuori dal carcere, per coloro che hanno commesso Il ricorso alle misure alternative alla detenzione in carcere e al reinserimento delle persone detenute attraverso il lavoro sono uno strumento valido, efficace, sicuro ed economicamente vantaggioso per attuare davvero l'articolo 27 della nostra Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Per contribuire a ridurre il sovraffollamento e migliorare così le condizioni di vita dei carcerati, potrebbe inoltre essere presa in considerazione la possibilità di consentire che gli extracomunitari che commettano reati possano scontare la pena nel Paese di origine

*(M5S)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi cittadini, prima di entrare nel merito del provvedimento permettetemi di fare tre o quattro considerazioni preliminari. luogo, questo decreto-legge non risolve affatto il problema della sovrappopolazione carceraria. Nella migliore delle ipotesi il Governo prevede l'uscita di non più di 3.000-4.000 condannati, a fronte di circa 20.000 esuberi totali rispetto alla capacità di accoglienza delle carceri italiane. Seconda considerazione. La stessa ministra della giustizia Cancellieri, invocando l'opportunità di un ulteriore - l'ennesimo e, aggiungo, malaugurato - provvedimento di amnistia o indulto per lenire il grave problema del sovraffollamento carcerario, ci ha indirettamente segnalato l'inefficacia complessiva di questo provvedimento, che affronta il problema senza risolverlo. Terza considerazione. Una parte importante del decreto-legge in materia di esecuzione della pena tratta un argomento che non ha nulla a che fare con l'esecuzione della pena: pena: l'attribuzione di nuovi compiti al Commissario straordinario di Governo per le infrastrutture carcerarie. La parola «straordinario» viene troppo spesso declinata da questo Governo. Si tratta di una scelta infelice che riporta alla mente, tra le altre cose, il ben noto scandalo della Protezione civile. In Italia, purtroppo, il ricorso alla straordinarietà degli interventi è una regola piuttosto che un'eccezione. Il sospetto è che possano essere create ad arte situazioni emergenziali per adottare decisioni in deroga alle regole. Quarta e ultima considerazione. La scelta del Governo di intervenire con decreto-legge certo non è giustificata dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in quanto questo provvedimento non affronta, se non in maniera marginale, il sovraffollamento carcerario. Questo decreto-legge scippa quest'Aula e il Parlamento tutto della funzione d'iniziativa e, quel che è peggio, della possibilità di un doveroso confronto con i cittadini su un tema che andrà a modificare sensibilmente il livello di sicurezza degli italiani e che avrebbe richiesto un dibattito di ben più ampio respiro nel nostro Paese. Forse non è un caso che ben 64 pagine di emendamenti siano stati resi disponibili solo la sera prima dell'arrivo in Aula di questo provvedimento, a voler sancire che l'opposizione non deve avere quel ruolo di controllore critico dell'attività della maggioranza che le spetterebbe di diritto. Avremmo voluto, gentili colleghi, un provvedimento molto diverso da questo per affrontare il problema del sovraffollamento nelle carceri: avremmo voluto, ad esempio, un piano per la messa in funzione delle numerose carceri presenti sul territorio che risultano ad oggi inutilizzate; avremmo voluto dei progetti per far lavorare i detenuti, che nella stragrande maggioranza restano chiusi in cella per la gran parte del giorno, ciò che favorisce naturalmente l'acuirsi delle tensioni; avremmo voluto un impegno straordinario del Governo - questo sì straordinario - per dare piena efficacia agli accordi bilaterali con agli altri Stati, che ci sono ma non funzionano al fine di consentire che sempre più extracomunitari detenuti possano scontare le loro pene nei Paesi di origine. Ma nulla di tutto questo è stato fatto. Al contrario, l'articolo 1 del decreto-legge in conversione stabilisce una possibile applicazione della liberazione anticipata e la possibilità per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione per dar modo al condannato di chiedere al tribunale di sorveglianza, da libero, una misura alternativa al carcere. L'articolo 2, sinteticamente, elimina le disposizioni restrittive concernenti le detenzioni domiciliari dei recidivi. L'articolo 3 consente al condannato tossicodipendente di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità

amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 3 dicembre 2012, integralmente richiamato dallo stesso. Al Commissario viene riconosciuto un aumento di organico, nonché la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato. A tale fine, va ricordato che le risorse affluenti alla gestione commissariale risultano fuori bilancio in quanto gestite a valere gestite a valere su una contabilità speciale di tesoreria. Le somme possono essere dunque gestite in deroga al principio tassativo di annualità, tipico della contabilità generale dello Stato. Non si vede però come, a dispetto della clausola di invarianza, queste risorse possano fronteggiare la proroga al 31 dicembre 2014 e le ulteriori funzioni dell'ufficio. Contraria alla normativa ordinaria è la possibilità di distacco e comando di pubblici dipendenti presso il Commissario, laddove si prevede che sia l'amministrazione di appartenenza a sostenere gli oneri per il trattamento fondamentale ed accessorio. Quanto alle nuove assunzioni a tempo determinato, esse non sono in linea con il dimezzamento del ricorso a tali figure contrattuali previsto dal decreto legge n. 78 del 2010. In generale, dunque, l'intero articolo 4 fa riferimento a un limite massimo di spesa la cui copertura è individuata in un capitolo che il Servizio bilancio del Senato sostiene di non avere individuato. Ne conseguono, per l'articolo 5, problemi di copertura finanziaria assai rilevanti, non adeguatamente sciolti dalla relazione tecnica, nonostante il fatto che la legge di contabilità, all'articolo 17, preveda che ogni clausola di invarianza sia debitamente dimostrata. In conclusione, il Movimento 5 Stelle, che ha più volte criticato il ricorso allo strumento delle gestioni commissariali straordinarie e derogatorie, intende impedire la proroga annuale e l'estensione dei poteri del Commissario straordinario per le carceri. Il Movimento Cinque Stelle propone, al contrario, di sopprimere il Commissariato straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e riattribuire le funzioni al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), peraltro già investito di tale funzione La *ratio* di tale proposta sta nella necessità di non ricorrere, come regola, alla straordinarietà degli interventi. Già nel 2008, infatti, venne nominato il Commissario straordinario, ma poi la legge n. 199 del 2010 e il decreto-legge n. 211 hanno introdotto ulteriori misure per ridurre il sovraffollamento. Nel 2012, a seguito della riduzione delle risorse disponibili, il piano straordinario è stato rimodulato, ma non sembra finora aver prodotto alcun risultato significativo, come dimostra la stessa esistenza di questo decreto.

in Commissione sanità abbiamo esaminato il disegno di legge in sede consultiva, ma nella consapevolezza e convinzione che le questioni sanitarie e, quindi, di nostra competenza non potevano essere esaminate se non in un'ottica parallela e trasversale alle questioni sociali, giuridiche e istituzionali. Per questo motivo abbiamo audito l'ANCI, il DAP e l'Istituto superiore di sanità penitenziaria ed i rappresentanti del tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria. Dopo tali audizioni, anche a seguito del parere espresso in Commissione e pur riconoscendo che il decreto‑legge oggetto di conversione rappresenta un passo avanti concreto per migliorare la situazione delle carceri italiane, situazione segnata da un sovraffollamento già ufficialmente condannato e sanzionato dal tribunale di Strasburgo e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in quanto si configura come una situazione insopportabile per un Paese civile, riteniamo che ci siano ancora molte cose da fare presto, puntualizzare

delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature in materia di sanità penitenziaria, la situazione delle carceri, dal punto di vista sanitario, rischia di diventare esplosiva. Dal febbraio 2009 è operativo presso la Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali il tavolo di consultazione permanente sull'attuazione del decreto

sedi di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Abbiamo, dunque, presentato un ordine del giorno nel quale si chiede al Governo un ulteriore impegno rispetto a quanto previsto dal disegno di legge di conversione per favorire un miglioramento dell'organizzazione dei servizi sanitari di base nell'ambito della sanità penitenziaria in conformità ai criteri di appropriatezza e alla necessità di assicurare la salute dei detenuti in un contesto di rete. Abbiamo chiesto al Governo di curare, per quanto di competenza e in collaborazione con le Regioni, che l'assistenza specialistica ambulatoriale sia conformata a criteri di razionalizzazione di domanda e offerta prevedendo presenze programmate in base alla valutazione epidemiologica delle patologie prevalenti; di assicurare che i detenuti sottoposti a un regime di media e alta sicurezza, che necessitano di assistenza continuativa in quanto affetti da patologie croniche, siano assistiti in istituti in grado di coniugare le esigenze di tutela della salute con quelle di sicurezza, attraverso la presenza di servizi sanitari con personale specializzato funzionanti nelle ventiquattrore; di istituire un organo di raccordo interistituzionale a livello centrale, preferibilmente in sede di Conferenza unificata, che possa costituire la sede dove concordare gli strumenti attuativi della legislazione intesa ad affrontare le problematiche della sanità penitenziaria in relazione alla più ampia questione dell'emergenza carcere. In ultimo, ma non per ultimo, chiediamo di monitorare attentamente e continuativamente le attività esecutive della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, adottando in maniera tempestiva ogni iniziativa necessaria ad evitare che si debba ricorrere nuovamente a provvedimenti di urgenza di proroga termini, ivi incluso l'esercizio dei poteri sostitutivi, *ex* articolo

si sia invertita o che, almeno, si sia tentato di invertire la tendenza che ha prodotto l'emanazione di una serie di leggi che hanno avuto come inevitabile conseguenza il riempimento a dismisura delle carceri italiane rendendo quello strumento straordinario che fu varato alcuni anni fa (cioè l'indulto) sostanzialmente insufficiente. Peraltro, dico subito che condividiamo anche alcune delle perplessità di queste ore dell'Unione delle camere penali rispetto al rischio

oggettivamente delicato, cioè il tema della recidiva reiterata e specifica. In ogni caso, noi pensiamo che invece questo debba essere il primo punto di partenza, se posso dire così,

e alla legge sull'immigrazione, che, a nostro avviso, sono la principale causa dal sovraffollamento, oltre ad avere introdotto nel nostro ordinamento principi giuridici che dal nostro punto di vista sono totalmente sbagliati. È per questo che, nel corso di questi giorni, siamo impegnati come Sinistra Ecologia Libertà a raccogliere le firme sui tre disegni di legge di iniziativa popolare per la giustizia e i diritti: quello che vuole introdurre modifiche alla legge sulla droga, depenalizzando il consumo e riducendo l'impatto penale, cioè rimodulando le pene e revisionando l'accesso ai programmi di recupero per i detenuti tossicodipendenti; quello per la legalità il rispetto della Costituzione nelle carceri, che chiede la conversione della pena nel caso in cui dovessero mancare i posti disponibili, modificando anche in questo caso la recidiva, il sistema dei benefici e l'accesso alle pene alternative; e quello, di cui abbiamo discusso spesso, la cui mancanza rappresenta a nostro avviso una gravissima anomalia del nostro sistema giuridico, relativo all'introduzione nel codice penale del reato di tortura, così come previsto dalle convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dal nostro Paese. Esattamente per le stesse ragioni vogliamo anche annunciare il nostro sostegno ad alcuni *referendum* radicali, in particolare quello relativo all'abrogazione del reato di clandestinità, che dal nostro punto di vista è un reato aberrante perché punisce una condizione anziché una condotta, e per eliminare anche quelle norme che incidono sulla precarizzazione dei lavoratori migranti. Insomma, per tutte queste ragioni che ho tentato di dire, guardiamo con favore a questi provvedimenti che si stanno portando avanti e anche a quelli che nelle Commissioni giustizia di Senato e Camera sono in corso di discussione in questi giorni e che sembrano voler andare finalmente verso una diversa idea di contrasto della delinquenza, cercando cioè di valorizzare quegli strumenti, alcuni dei quali, peraltro, già presenti nella legislazione minorile (è il caso, per esempio, della messa in prova, che è allo studio delle Commissioni parlamentari), capaci di interrompere quella spirale cosiddetta delle porte girevoli, la repressione dell'attività delinquenziale attraverso il carcere non riesce a compiere né la rieducazione del condannato, prevista della nostra Costituzione, e nemmeno la sua sottrazione, per l'appunto, dalla spirale delinquenziale. Per queste ragioni noi guardiamo con favore allo sforzo fatto dal Governo, che, pur senza stravolgere, naturalmente, l'ordinamento attuale, intende però realizzare un alleggerimento del nostro sistema penitenziario, favorendo l'adozione di meccanismi di decarcerizzazione in relazione a persone considerate di non elevata pericolosità, ferma restando, naturalmente, la necessità dell'ingresso in carcere di quei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale, fattispecie tra cui - abbiamo preparato su questo anche un emendamento - rientra a nostro avviso, differentemente dal testo originario del Governo, certamente l'incendio boschivo. Consideriamo e condividiamo in particolare tutti quegli istituti che premiano con una riduzione di pena il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere, sia l'estensione della misura degli arresti domiciliari, sia l'ampliamento della possibilità che ha il giudice di ricorrere a misure alternative al carcere, a partire dai lavori di pubblica utilità. Ci sembra anche - e ne parleremo più diffusamente più tardi in sede di dichiarazione di voto - che sia questa ispirazione di fondo a rendere questo decreto condivisibile, vista la nostra convinzione, da molti anni a questa parte, che le leggi recentemente introdotte, invece, siano andate in un'altra direzione. Si pensi ad una legge mai sufficientemente criticata come la *ex* Cirielli del 2005, dal nostro punto di vista garantista ai limiti dell'indulgenza verso alcune particolari categorie di persone e di reati e invece giustizialista fino in fondo e incapace di produrre risultati concreti in particolare verso i recidivi, dei quali si immaginava di infierire, come tra l'altro è stato recentemente e autorevolmente ricordato, con un meccanismo simile (forse qualcuno di voi lo ricorderà) a quello che vigeva un tempo in alcuni Stati americani, in particolare, per esempio, nella California, dove l'aver commesso tre reati consecutivi nella propria vita, indipendentemente dal tempo che separava un reato dall'altro o anche dalla tipologia di reato, determinava pene severissime, fino addirittura all'ergastolo. A seguito dell'approvazione di quella legge e con il combinato disposto delle leggi sull'immigrazione e sulle droghe, la popolazione carceraria è aumentata nel nostro Paese in pochi anni di più di un terzo, dai circa 40.000 detenuti ai circa 60.000 attuali, in una condizione come quella italiana in cui la capienza tollerata potrebbe arrivare al massimo a 45.000 persone. oltre al lavoro importante fatto in questi anni dal difensore civico e anche dalle associazioni che da anni si battono meritoriamente per i diritti della popolazione detenuta, ha determinato, com'è stato ricordato anche stamattina in Aula, la reazione dell'Europa e in particolare della Corte europea dei diritti umani rispetto alle centinaia di ricorsi che sono stati presentati. Com'è noto, la Corte di Strasburgo non si è limitata ad una declaratoria di condanna nei confronti dell'Italia, ma ha emesso una vera e propria sentenza pilota, con la quale è stato assegnato al nostro Stato un termine pari ad un anno entro il quale occorrerà procedere all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell'articolo 3

a preferire la strada dell'assegnazione di un termine in luogo di quella, peraltro inutile agli effetti pratici, di una statuizione di condanna a carico dell'Italia. Com'è stato autorevolmente ricordato, a distanza di tre anni dalla sentenza Sulejmanovic l'Italia, con la sentenza pilota Torreggiani, è dunque tornata al centro delle attenzioni della Corte di Strasburgo

così da determinare un sovraffollamento del 150 per cento e gli interventi che furono previsti all'epoca nell'ambito del piano carceri che fu immaginato per contenere il fenomeno, si sono finora rivelati del tutto privi di efficacia nel contrastare appunto il problema del sovraffollamento, tant'è vero che due anni dopo, nel 2012, la popolazione carceraria era diminuita, rispetto al 2010, di sole 1.500 persone,

dicendo che per noi l'unico vero motivo di rammarico è che il Governo e il Parlamento sono intervenuti su questa materia più sulla base di una normativa stringente europea che sulla base di un proprio convincimento profondo. Questo ci dispiace, eppure pensiamo che questo decreto possa essere, se non certamente la soluzione, almeno un primo passo per contrastare una situazione eccezionale che richiede strumenti anch'essi eccezionali, a partire, a nostro avviso, anche dalla stessa amnistia, di cui discuteremo in altre sedi e in altre occasioni.

dai quali il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati non si possono più esimere. Parto Parto sempre dall'ultimo commento del collega che parlava della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha più volte accolto i ricorsi dei proponenti, specialmente per quanto attiene ai temi legati all'amministrazione della giustizia, ad esempio per quanto riguarda i termini di durata dei processi. Tengo a precisare che questo costa all'Italia - signor Sottosegretario, se lo appunti - 31 miliardi di euro. Questa mala giustizia - signor Sottosegretario, lo dica al suo ministro Cancellieri

che sono veri e propri*lager*. Io dimostrerò alla fine del mio intervento che c'è poca differenza tra come stavano gli internati nei campi di concentramento nell'ultima guerra mondiale e quello che succede qui. Che differenza c'è tra le nostri carceri, quelle di Auschwitz o quelle dei Piombi della Repubblica veneziana? Il collega faceva riferimento alla sentenza Torreggiani ed altri in Italia, che è una delle ultime sentenze in materia. Per ragioni dovute al sovraffollamento carcerario e, più in generale, alle condizioni nelle quali i detenuti ricorrenti hanno affrontato la detenzione, la Corte ha riscontrato, signor Sottosegretario, una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà.

La Corte, infatti, ha accertato che: «i ricorrenti abbiano subito un danno morale certo» per le cattive condizioni in cui hanno affrontato la detenzione: come ad Auschwitz, come nei Piombi di Venezia. La Corte ha anche disposto che l'Italia dovrà «istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi ed idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario». La mala giustizia ci costa, oltre ai 31 miliardi di euro della lentezza, un punto di PIL, che, ricordo per chi non è avvezzo a fare i conti,

un signore suicidato a domicilio, perché gli si doveva far fare il carcere: Raul Gardini. Non si è suicidato, l'hanno suicidato, perché avevano paura che parlasse della *lobby* dei giornalisti economici, che pilotavano, ovviamente, le varie ripartizioni dei mercati, da una parte o dall'altra,

al Mugello e poi Ministro dei lavori pubblici. Dopodiché, lo hanno apparentato, al posto dei socialisti, nel 2008, con l'Italia dei Valori, lasciando Boselli e i socialisti fuori da quell'apparentamento. Certo, ciò è costato a quel partito, che ha dovuto pagare per anni, anni, ovviamente disobbligarsi e quindi aiutarlo in tutti i modi per non avere subito il trattamento che meritava a quel tempo.

il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, con l'adozione della raccomandazione Rec R(99)22 ha invitato gli Stati e l'Italia ad esortare procuratori e giudici, signor Sottosegretario, a ricorrere quanto più a ricorrere quanto più possibile a misure alternative alla detenzione e a limitare il ricorso alla carcerazione, e questo sia per motivi motivi legati ai diritti che per questioni attinenti meramente all'emergenza carceraria: non per l'emergenza, dice questa raccomandazione (e voi sapete che le raccomandazioni sono legge per noi), non per il sovraffollamento, ma per i diritti La suddetta raccomandazione evidenzia che «l'ampliamento del parco penitenziario dovrebbe essere piuttosto una misura eccezionale in quanto, in generale, non è adatta ad offrire una soluzione duratura al problema del sovraffollamento»; e ancora, testualmente, dice: «È opportuno prevedere un insieme appropriato di sanzioni e di misure applicate nella comunità, eventualmente graduate in termini di gravità»; inoltre, testualmente dice, signor Sottosegretario: «Gli Stati membri dovrebbero esaminare l'opportunità di depenalizzare alcuni tipi di delitti o di riqualificarli in modo da evitare che essi richiedano l'applicazione di pene privative della libertà». Il provvedimento in esame si pone, dunque, in scia con le direttrici europee che abbiamo sottoscritto come Stato membro e che non possiamo quindi ignorare. Non possiamo ignorare perché è giusto prendere in considerazione le due donne kazake, la madre e la figlia, che hanno subito oltraggio

Inoltre, il decreto interviene in via incidentale anche sull'annosa problematica relativa alla certezza della pena che, purtroppo, spesso risulta inapplicabile a causa di *deficit* strutturali o per una legislazione inadeguata perché non aggiornata. pena occorrono misure (e questo decreto ne contiene alcune) in grado di assicurarne l'effettività, senza al contempo violare i diritti garantiti dalla nostra Costituzione, dai trattati, dalle intese e dalle convenzioni europee. Non dimentichiamo che, oltre alla sua funzione meramente punitiva, la sanzione vuole assolvere anche al compito di rieducare e riabilitare il reo che, comunque - è bene evidenziarlo - mantiene sempre alcuni dei diritti fondamentali che la Costituzione gli garantisce.

i diritti umani, a qualsiasi grado e a qualsiasi livello. Così pure quanti sono sottoposti a misure limitative della libertà personale devono vedersi assicurate le previsioni della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario. Se lo stato degli istituti di

per questo la ringrazio, e credo - e spero - che il *racket* dei magistrati non le abbia fatto cambiare il parere, altrimenti dovrei lanciarle, in mezzo a quest'Aula il guanto di sfida, perché noi socialisti non arretriamo di fronte a nessuno: abbiamo liberato l'Italia dai fascisti e siamo in grado di liberarla anche dai giudici cattocomunisti. Tutti i servizi e le attività in carcere sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per cui l'istituto è stato progettato: la qualità complessiva della vita in un un istituto si abbassa anche in maniera significativa; inoltre il livello di sovraffollamento in carcere, o in una parte particolare di esso, potrebbe essere tale da essere inumano

che non consenta l'effettiva riabilitazione e rieducazione del condannato per inidoneità strutturali e igienico‑sanitarie o, infine, che esponga il detenuto, per le medesime cause, a contrarre affezioni psico-fisiche o malattie infettivo-diffusive. Chiunque permetta questo, in base all'articolo 608 del codice

che mettono in carcere le persone in queste condizioni: lo dice il nostro codice penale. Perché allora non si applica? Si tratta di una casta di persone che guadagna di più, hanno il doppio di mesi di ferie, fanno una o due sentenze l'anno e non pagano per gli errori che fanno, anche volutamente,

Signor Presidente, in questa fase della discussione generale svolgerò soltanto alcune riflessioni di carattere generale perché, per quanto riguarda il merito, *in parte qua* ero già intervenuto in sede iniziale di esame della questione pregiudiziale di costituzionalità.

questa sede quasi da ricordare il paradosso secondo cui bisognerebbe intervenire con decreto-legge per sistemare il processo penale e tutto il sistema penale che sta andando a scatafascio. La situazione è vicina al fallimento, per cui avrebbe bisogno di interventi radicali

sono profondamente convinto della necessità di arrivare a modifiche profonde del nostro codice penale, il quale - ricordiamolo ancora - nella sua impostazione originaria risale al 1930,

Cito, ad esempio, la materia della depenalizzazione e la necessità di rivedere certe norme criminogene, la persistenza degli effetti deleteri delle leggi Bossi-Fini e Fini-Giovanardi. Oltre ad intervenire sul sistema penale, reputo opportuno - come abbiamo proposto, ed esistono già proposte in tal senso in sede di Commissione giustizia del Senato - intervenire sul codice di procedura penale, ossia su quelle misure che conducono alla custodia cautelare e al carcere.

se si dovesse decidere di intervenire su tutti questi aspetti del sistema penale nel suo insieme, alla fine si potrebbe anche ragionare in materia di indulto, come qualche senatore ha proposto; non certo in questo momento momento e in questa situazione: non ci troviamo nelle condizioni di intervenire con misure così radicali e pesanti che potrebbero procurare solo danni rispetto a quella che sarebbe l'intenzione. dalla misura dell'indulto adottata nel 2006, c'è stato un lieve sospiro di sollievo per qualche mese, ma poi la situazione è tornata ad essere quella di prima. Pertanto, se si vuole intervenire nell'ambito del

corso del mio primo intervento ho parlato della necessità di pensare di risolvere la questione del sovraffollamento penitenziario. Si tratta, in particolar modo, di un profilo

profilo, a mio modo di vedere, si tratta di una misura ancora timida, ancora limitata, perché essa potrà dare sollievo in determinate situazioni ma certamente non risolverà il problema del sistema penale nel suo insieme. È indubbio che questo decreto‑legge avrà un effetto deflattivo sulla popolazione carceraria e consentirà, per così dire, di riequilibrare il sistema esecutivo della pena, eliminando in particolar modo almeno una parte di quegli automatismi così rigidi e privi di significato che erano stati posti nell'ottica di una difesa sociale, peraltro male interpretata. Per altri meccanismi, che pur rimangono,

che non destano allarme sociale e che sono determinate più che altro da un far scorrere le acque senza intervenire decisamente, così come determinati casi meriterebbero.

questo intervento normativo si pone in termini di urgenza per fronteggiare un caso drammatico di sovraffollamento carcerario derivante dall'inadeguatezza delle strutture e anche, forse, da una insistenza eccessiva nell'applicare, quasi esclusivamente o prevalentemente, sanzioni detentive in luogo di altre che potrebbero essere sviluppate. già dall'articolo 1 questo provvedimento interviene modificando gli articoli del codice di procedura penale, consentendo di allargare l'ambito di applicazione degli arresti domiciliari e anche della sospensione degli ordini di esecuzione di pene detentive. Quindi, la *ratio* di questa normativa è evidente: un effetto deflattivo certamente raggiungibile con questo intervento. Come è già stato rappresentato dai colleghi che mi hanno preceduto, e ribadito in ultimo dal senatore Casson, esistono delle rigidità

per una regola (faccio un esempio per tutti) chi ha riportato già delle condanne, indipendentemente dalla gravità o dal tipo di reato che ha consumato, per il solo fatto di trovarsi in questa condizione, non può essere ammesso ad usufruire di questa normativa L'articolo 2 riguarda l'ordinamento penitenziario, e anche in questo caso sono stati previsti ampliamenti della possibilità di applicare la detenzione domiciliare;

L'articolo 4 amplia lodevolmente gli interventi che possono essere svolti dal commissario

L'articolo 6 riguarda la decorrenza - è un fatto quasi ordinario

significato per rappresentare - appunto - la tensione del sistema detentivo italiano sono evidenti; alcuni colleghi li hanno già citati, ma giova ripeterli: nel 2010 vi

ci spiace ammetterlo in quest'Aula, ma è un dato di realtà - la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all'adozione di misure necessarie a porvi rimedio. Spunti interessanti per caratterizzare questo orientamento, oltre alla già citata sentenza, si trovano anche nella Raccomandazione dei principi base che i Governi degli Stati membri devono adottare in materia di sovraffollamento della carceri e di infiltrazione carceraria,

Gli Stati membri dovrebbero esaminare - cito il punto - l'opportunità di depenalizzare alcuni tipi di delitti e riqualificarli, in modo da evitare l'applicazione di pene privative della libertà. Quindi, coerentemente con questi principi, che ci richiamano alla civiltà giuridica del nostro Paese, insieme alla nostra appartenenza all'Unione europea,

C'è un problema reale, un problema vero, ossia il sovraffollamento nelle carceri: non è una novità, non è una questione che ci troviamo ad affrontare adesso perché è emersa da qualche giorno o da qualche settimana; è un problema decennale, è un problema che viene dal passato, per risolvere il quale pochissime cose sono state fatte,

altrimenti non andiamo da nessuna parte e seminiamo solo paura; altrimenti sono solo espedienti.

a seguito del gesto che sappiamo: è uno di quegli 8.000 sindaci (che ho seguito molto modestamente da Sottosegretario con delega agli enti locali) uno di quegli 8.000 eroi che ci sono sul territorio,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra è la tragedia di un Paese che non è serio: in quest'Aula si presenta un decreto-legge con cui si commissaria il Ministero della giustizia per compiti istituzionali. Non si sta parlando di interventi straordinari, ma semplicemente di gestire i flussi di ingresso e di uscita dei detenuti e di un piano carceri: e per questo si prevede un Commissario straordinario?

onorevoli colleghi, che si vuole utilizzare lo strumento del commissario straordinario, come è stato ben detto dai miei colleghi. Nelle norme che lo prevedono c'è un'intera pagina di deroghe alle norme comunitarie sugli appalti: si vuole fare entrare la mafia e la corruzione anche nel piano carceri. Questa è una vergogna indicibile! È una vergogna indicibile l'uso dei commissari straordinari! Sappiamo come sono andati a finire negli anni: non ce n'è uno che non sia finito davanti alla magistratura. Lo sappiamo bene perché il problema non è

C'è un'altra ipocrisia, cari colleghi. Un paio di giorni fa, in violazione della Costituzione, non abbiamo sanzionato l'operato di un Ministro e del suo Ministero, come previsto all'articolo 95 della Costituzione, che ha compiuto un atto di barbarie contro una donna e una bambina. In quest'Aula ci sono tanti tanti che si strappano le vesti e fanno interventi strappalacrime perché sono preoccupati dei detenuti: con quale coraggio li fanno, dopo aver ratificato l'operato del Ministro la scorsa settimana?

un atto di grave slealtà nei confronti del Parlamento e dell'opposizione, e come tale sarà trattato dal Movimento 5 Stelle nelle prossime sedute.

avanti un altro tipo di opposizione: quella a cui ci avete costretto per fare il nostro dovere nei confronti dei cittadini.

prendo la parola senza nascondere soddisfazione e ottimismo per l'argomento di cui parliamo quest'oggi: la conversione in legge del decreto-legge in materia di esecuzione della pena e di emergenza nelle carceri italiane. Giungiamo a questa fase dopo un intenso e proficuo dibattito e lavoro in sede di Commissione giustizia, dove il problema del sovraffollamento carcerario è stato certamente uno dei temi che ha caratterizzato la legislatura. L'emergenza del problema in oggetto, oltre che essere testimoniata dai fatti che quotidianamente la cronaca ci descrive, si rileva da seri e dettagliati dati in materia. Questa gravità, inoltre, è sottolineata dalle continue condanne dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea dei diritti dell'uomo. Strasburgo ha evidenziato l'assenza di un piano di edilizia carceraria, stigmatizzando la politica penitenziaria italiana e l'assenza di opportune norme di depenalizzazione e misure alternative. Per il sovraffollamento delle carceri il nostro Paese è al terzo posto in Europa; davanti a noi ci sono solo Serbia e Grecia. Si tratta di una realtà che pone i nostri strumenti detentivi al limite della legalità, dove perdura una situazione divergente dalle regole poiché non si è in grado di garantire, nella maggior parte dei casi, quanto previsto dalle normative vigenti e dal regolamento penitenziario. Secondo il Ministero della giustizia, dopo l'indulto del 2006, la popolazione carceraria passò da 61.264 detenuti nel giugno a 39.005 dello stesso anno; negli anni successivi, dopo un rapido ritorno alla situazione pre-indulto, le presenze aumentarono nuovamente toccando, nel 2010, le 67.961 unità. Negli anni 2011-2012, dopo un miglioramento della capienza degli istituti e una lieve diminuzione della popolazione carceraria, i dati più recenti hanno registrato nuovamente un aumento: nel febbraio 2013, infatti, erano presenti nelle carceri italiane 65.906 detenuti. I dati statistici, con le loro cifre, rappresentano anche il paradigma della civiltà democratica di ogni Paese e, in tal senso, i nostri dati non ci fanno certo essere orgogliosi. Per far fronte a questo grave problema di ordine sociale per il Paese, nel 2010 il Governo, dopo la nomina nel 2008 di un commissario straordinario, deliberò un piano straordinario basato su un'articolata serie di interventi, prevalentemente di edilizia penitenziaria, dichiarando lo stato di emergenza nazionale. Il piano carceri, che avrebbe dovuto creare circa 18.000 nuovi posti detentivi entro il 2012, era articolato in quattro filoni di interventi, alla cui base vi era appunto la dichiarazione dello stato di emergenza carceraria. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che affrontiamo costituisce un argomento di larga attualità che interpella la coscienza civile e politica. Oltre ai dati succitati, basta aggiungerne altri per comprendere ancor più che ci si trova dinanzi a un'emergenza che rendeva necessarie immediate e improrogabili risposte, concrete quanto efficaci. Gli allarmanti segnali di questo disagio sono continuamente forniti anche dalle crescenti proteste dei detenuti, con migliaia di scioperi della fame e gesti di autolesionismo, fino ai numerosi casi di suicidio: troppi. troppi. Al sovraffollamento si aggiungono le scarse spese per l'assistenza psicologica e le attività culturali. Anche il personale della Polizia penitenziaria è sotto organico. Questa realtà si scontra con la garanzia costituzionale della funzione rieducativa della pena, tanto che oltre il 65 per cento degli ex detenuti torna a delinquere. Un elemento particolarmente significativo che ci fa riflettere è quello di una popolazione carceraria formata per due terzi da immigrati e tossicodipendenti; si tratta di fasce deboli dell'ormai variegata società italiana e persone verso cui un atteggiamento repressivo si è rivelato per lo più un danno sociale. In tale circostanza, il piano carceri, che prevede la costruzione di nuove strutture, va sicuramente accompagnato da un moderno e diverso strumento di recupero sociale dei detenuti. dei detenuti. L'alternativa al carcere non significa affatto non scontare la condanna, ma sostituire la pene detentiva con un recupero della persona tramite servizi di utilità sociale, così come avviene nei sistemi giuridici di tradizione anglosassone. l'obiettivo della classe politica dirigente non può e non deve essere riempire le prigioni, ma svuotarle e non solo attraverso le amnistie, di cui si è abusato nel passato, essere fatte anche oggi, visto lo stato di emergenza, unitamente, come è stato ripetuto, alle riforme di tipo sostanziale e processuale; questo se tutte le forze politiche fossero concordi, al di là dell'impopolarità di tale misura) ma anche attraverso un piano di depenalizzazione dei reati minori, (nel nostro ordinamento vi sono moltissime fattispecie di reato) cioè, l'eliminazione dai codici di quei reati che destano scarso allarme sociale. Insomma, cambiare la legislazione in materia è adesso un obbligo morale e proprio in tale direzione va il decreto-legge che sarà convertito in legge. Come ho prima accennato, nelle fasi di emergenza anche l'amnistia può essere un'efficace soluzione al sovraffollamento delle carceri, ma il problema va risolto radicalmente alla base. Ribadisco che oltre alle misure alternative alla detenzione carceraria, la depenalizzazione costituisce la soluzione migliore al problema in questione. Mi piace sottolineare il principio per cui uno Stato moderno deve essere rigoroso nell'applicazione della certezza della pena e, allo stesso tempo, rispettoso dei diritti che tutelano la dignità della persona, come dell'intera società civile. Sono certo che la depenalizzazione, se ben applicata, risponderebbe appieno a tali principi. Chiaramente, il principio dell'effettività della pena non può essere eluso, ma va sottolineata la funzione rieducativa della pena, la stretta relazione tra rieducazione e bisogno di sicurezza. Dopo essere stata condannata una persona viene consegnata a un luogo che è un contesto dove convivono numerose altre persone, compresi coloro che sono predisposti alla loro custodia, dove si avvia il percorso del trattamento rieducativo. In questa fase delicata lo Stato non può più ridurre la sua politica ad una mera azione segregativa-assistenzialistica; infatti, in questa fase il carcere dovrebbe essere l'*extrema ratio* dell'intervento punitivo. Già Francesco Carnelutti affermava che: «Il processo penale avrebbe fallito il suo scopo se anche con l'irrogazione della giusta pena non si fosse raggiunto l'obiettivo del riabbraccio ultimo tra la società e il reo». Lo Stato dovrebbe quindi intervenire con modalità diverse, con cui anche soggetti pubblici e privati, o associazioni, possono operare per realizzare una sicurezza integrata, dove si ipoteca l'inserimento sociale del condannato e si tutelano i cittadini e il territorio dalla devianza di ritorno, cioè dalla recidiva. Le carceri ci fanno pensare alle città invisibili di cui scriveva Italo Calvino. In effetti, il pensiero comune è quello di considerarle fuori dalla società; invece, a me piace pensare al carcere come parte della società, come qualcosa che si pone non al di fuori della città, ma dentro la città, in un rapporto integrato e costruttivo con il tessuto sociale in cui esso insiste, dove i detenuti possono essere impegnati in lavori socialmente utili. Un illustre sociologo, Loïc Wacquant, ha evidenziato come i detenuti che non svolgono alcuna attività vivono quella condizione che si definisce di neutralizzazione dei corpi, dove essi sono posteggiati nel modo peggiore; come in «Resurrezione» di Tolstoj, anche questa è un'umanità sconosciuta, che fa parte anch'essa di questo mondo. Ricordo qui il magistrato di sorveglianza di Lecce che di recente ha qualificato certi trattamenti carcerari dovuti al sovraffollamento, degradanti e lesivi per la dignità umana. In tali aberranti circostanze si passa da uno Stato sociale a uno Stato penale, ed ecco che ribadisco ancora come il carcere rappresenta un indice del grado di civiltà di un Paese. In sostanza, il carcere-servizio pubblico deve essere un luogo che produce sicurezza collettiva nel rispetto della dignità umana dei detenuti. Sull'argomento, quindi, sarebbe necessario avviare una riflessione per ripensare ai processi brevi e alla certezza della pena, fornendo migliori strumenti e maggiori risorse. Sottolineando come il decreto-legge per la riforma del sistema carcerario si offre come uno strumento indispensabile e, per certi versi, decisivo ricordo che esso rappresenta innanzitutto un eccezionale cambiamento culturale, un orientamento nuovo, ma ancora incompiuto. Oggi la punizione prevale sul trattamento e il tempo del carcere diventa un tempo vuoto, senza opportunità di prospettive e di senso. Una riflessione si impone con obiettività e senza alcun preconcetto. Non si può continuare a riempire le carceri senza fare un ragionamento sul senso della pena. Senza voler mettere in discussione il principio di legalità si possono mutare o rivedere gli istituti già esistenti. A mio avviso, non abbiamo bisogno di nuove carceri, ma che i fondi destinati a tale scopo vengano usati per creare posti di lavoro per detenuti ed ex detenuti. Nella società vi è oggi una forte domanda di sicurezza ed in tale situazione le risposte devono nascere prioritariamente già dal carcere. In tale sede occorre cominciare ad operare per un reinserimento sociale, così da dare risposte concrete anche ai cittadini. Pertanto, è auspicabile che il Parlamento e le forze politiche continuino ad operare e cooperare in tale direzione per la ricomposizione di una realtà troppo a lungo disgregata, trascurata, e quindi fallimentare. Ciò per ricondurre la situazione nel contesto della vita democratica, e quindi civile, del nostro Paese.

a inizio gennaio - è bene ricordare da dove parte il percorso che ci porta qui - la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia, con la sentenza Torreggiani ed altri, per avere sottoposto 7 detenuti a trattamenti inumani e degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Erano incarcerati tra Busto Arsizio e Piacenza in uno spazio di tre metri quadrati a testa, meno dei quattro metri quadrati stabiliti come limite minimo dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Si è trattato, come è stato ricordato prima, di una sentenza pilota: una sorta di preavviso a mettersi in regola con le prescrizioni stabilite prima che si dia corso ad altre più pesanti sanzioni. Accanto a questo, lo stesso Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa aveva chiesto, attraverso numerose raccomandazioni, di ricorrere maggiormente a misure alternative alla detenzione e di considerare la privazione della libertà come l'estrema sanzione da riservare, come recita la raccomandazione n. 22 del 1999, ai casi in cui la gravità del reato è tale da rendere qualunque altra misura o sanzione manifestamente inadeguata. Non è così che viene utilizzata la pena carceraria in Italia. Oggi, la popolazione carceraria ammonta a più di 65.000 unità, a fronte di una capienza di 45.500 posti;

Le persone sottoposte a esecuzione penale esterna al carcere nel 2012 erano meno di 20.000: meno della metà di quanti erano sottoposti al medesimo trattamento dieci anni prima. all'esame, quindi, si mettono in campo alcune misure di alleggerimento della pressione demografica carceraria e contemporaneamente si cerca di avvicinare il sistema detentivo italiano a quella idea che ne aveva il nostro Cesare Beccaria: un luogo in cui la certezza della pena, e non la sua crudeltà, sia da deterrente ad altri delitti. Si salvaguardano i percorsi trattamentali per l'altissima percentuale di condannati tossicodipendenti; si limitano i casi delle cosiddette porte scorrevoli, le costosissime, e spesso inutili, permanenze in carcere per pochi giorni; si agevola la detenzione domiciliare delle mamme, in certi casi dei padri, con bambini piccoli. Insomma, si mettono in campo misure deflattive che hanno anche l'obiettivo di rendere un po' più umana l'applicazione della pena. Ma questo è un passo. Altre norme attendono di essere approvate per restituire alle carceri italiane il profilo di luoghi di rieducazione, e non di violazione della dignità umana: la modifica della legge sugli stupefacenti; l'introduzione del reato di tortura; la revisione delle norme sull'immigrazione, con l'abolizione del reato di clandestinità; l'istituzione del garante dei detenuti. garante dei detenuti. Insieme a queste misure, sarà importante recepire al più presto la direttiva europea n. 29 del 2012 su diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, perché uno dei peggiori effetti collaterali del malfunzionamento della giustizia italiana è la contrapposizione, frequente e in sé immotivata,

un sistema di esecuzione delle pene umano e insieme affidabile. Tanto più giuste sono le pene, scriveva Beccaria, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza e maggiore è la libertà che il sovrano conserva ai suoi sudditi:

Con un ultimo gesto di grande generosità, come lei voleva, la famiglia ha donato alcuni organi affinché altre persone abbiano nuova speranza di vita. Signor Presidente, confido nella sua sensibilità perché lei sappia trovare un momento per un minuto di silenzio in un'Aula magari meno vuota. Si tratta, infatti, di una sindaca che muore, ma non per cause accidentali. Come sapete, venti giorni fa un vigile del suo Comune, un omuncolo sospeso dal suo ufficio per truffa e peculato nell'esercizio delle sue funzioni, aveva sparato a lei e al vice sindaco durante il momento di ricevimento dei cittadini. Il vice sindaco è vivo, per fortuna. Laura no, lei non ce l'ha fatta. Noi che la conoscevamo abbiamo letto con grande rispetto e partecipazione le condoglianze delle più alte cariche dello Stato, quelle del nostro partito e di altri che sono intervenuti, che ricordano l'amministratrice capace, onesta e integerrima, ma sempre aperta ai bisogni dei suoi concittadini, che proprio quel giorno fatale, come di consueto, incontrava nel suo ufficio, senza timore per intimidazioni di sorta, che pure aveva ricevuto. Apprezziamo il ricordo della sua competenza, frutto di una gavetta che viene da lontano e di autentiche capacità: consigliera comunale, provinciale, assessora, vice sindaca e sindaca. Sappiamo della donna impegnata, presidente del PD provinciale, responsabile delle donne e per le donne, alle cui battaglie ha iniziato tante di noi, che devono anche a lei l'essere qui, nel luogo in cui la democrazia deve crescere e compiersi. So che vorrebbe fosse ricordata, altresì, come donna antifascista, convinta e fedele alla Costituzione. Oggi, però, lasciate che quest'Aula, che nel tempo ha sentito ben altri discorsi, declamati da persone di levatura assai maggiore della mia, ascolti parole povere e semplici. Lasciate che vi parli di un sorriso, incastonato tra due occhi azzurri e una massa di capelli biondi: quel sorriso di donna incantava, avvinceva, ma soprattutto comunicava. Poteva non parlare, Laura, ma sapevi comunque cosa provava. Potevi parlarle e sapevi da quel sorriso che ti ascoltava e cosa pensava. Si parla di fatalità, si parla di follia, come se fosse un incidente di percorso tra altri, che tra breve sarà dimenticato, un momento estremo in tempi difficili, come sentivo ieri in televisione, cercando di non sentire; come se la continua violenza verbale l'antipolitica militante, anche paludata da accademia o da neutrale servizio mediatico al servizio del cittadino, prive di analisi e attente quanto mai alle curve dei sondaggi, non avessero responsabilità alcuna. A chi fa comodo far di tutta l'erba un fascio? *Cui prodest*, si direbbe? Chi vuole ottenere qualcosa da tutto questo? Attendiamo risposte e proveremo a darle anche noi. Vuoi mai vedere che l'incidente di percorso è proprio quel sorriso determinato e ironico, tenero e combattivo che chi l'amava ha perso per sempre? Non lo permetteremo, Laura. Continueremo da dove hai lasciato. Partiremo da quella sera sul femminicidio, pochi giorni prima che ti rincorressero per spararti e ti raggiungessero dove ti eri rannicchiata - come mi hai detto - incredula prima ancora che impaurita, per tornare a spararti ancora e ancora. Lascia che oggi piangiamo con tuo marito Pino e i tuoi figli Massimo e Alessia. Lascia che la rabbia contro chi ti ha fatto questo gridi forte. Lasciaci consapevoli che non ci lascerai mai. Dovunque tu sia, sorridi: chi ha avuto la fortuna della tua confidenza saprà vederlo e riconoscerlo quel sorriso, ovunque giochi a nascondersi. Ciao, tesoro caro, amica e sorella. Ciao, sindaca. Da quest'Aula un abbraccio e una lacrima, che rimane nel cuore e non si asciugherà mai, per tutta la vita. Costruiremo per te un ricordo indelebile sul nostro territorio. Noi, le donne, le tue amiche, quelle che sono sempre state le tue sorelle, quelle che tu hai guidato in questo passaggio. Ciao, Laura. Ciao, tesoro mio. Un abbraccio.

Ho già espresso ieri il mio cordoglio ai familiari per questa perdita, a nome mio e dell'Assemblea. Invito ora tutti a osservare un momento di raccoglimento e di silenzio.

stanno proprio a Sud, nell'isola di Pantelleria. Tutti la conosciamo: un posto dove madre natura si è impegnata un po' di più, dove è riuscita a coniugare la terra con il mare, dove fa andare d'accordo e d'amore il fuoco con l'acqua, dove si può apprezzare un lago sul cratere di un vecchio vulcano. È un posto incantevole. Spesso però succede che, dove magari madre natura mette più impegno, l'uomo ce ne mette altrettanto per rendere meno vivibile

per le avverse condizioni meteo-marine, le navi o non partono proprio da Trapani o rimangono attraccate a Pantelleria. Le donne che devono che devono partorire ricevono un'assistenza fino alla trentaduesima settimana; arrivate alla trentaduesima settimana, il ginecologo di turno a Pantelleria invita

con la nave, ma ci vogliono ben sei ore. Allora, questo grido di allarme, questo mio intervento che vuol dare voce, signor Presidente, cari colleghi, ai cittadini panteschi,

lì dove vive, a ridare dignità ai padri che vogliono veder nascere il proprio figlio nell'isola in cui vivono. Per questo preannuncio che presenterò un'interrogazione urgente che sottoporrò alla sua attenzione, signor Presidente. dopo tre anni di lavoro la procura di Lucca ha rinviato a giudizio 42 imputati - 33 persone fisiche e 9 società - nell'ambito dell'inchiesta per il disastro ferroviario di Viareggio il più grave mai accaduto in Italia. A patire dal 13 novembre prossimo gli imputati dovranno comparire davanti al giudice per difendersi dai reati contestati: disastro ferroviario colposo, incendio colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime, oltre che, per alcuni, violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Sul banco degli imputati ci sono i vertici delle Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato del gruppo, Mauro Moretti, e gli amministratori

fatta dalla commissione di indagine ministeriale e dalla Direzione generale per le investigazioni ferroviarie del Ministero dei trasporti. Secondo notizie di stampa, nel corso dell'udienza preliminare, un avvocato della difesa avrebbe anticipato che il rinvio a giudizio dei vertici di Ferrovie dello Stato non inciderà in alcun modo sugli incarichi ricoperti da amministratori delegati e dirigenti coinvolti, ed è ciò che potrebbe verificarsi proprio il 25 luglio prossimo nell'assemblea del gruppo Ferrovie dello Stato, chiamata, tra l'altro, a decidere in merito al rinnovo del mandato - il terzo - di Mauro Moretti come amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato.

ieri, presso la ex Golden Lady di Gissi, in Abruzzo, i lavoratori tutti hanno presidiato la fabbrica per evitare che la stessa venisse smembrata con l'allontanamento o la rimozione dei macchinari. Mi sento vicino fisicamente, oltre che idealmente, a loro. Con questo intervento in Aula cerco di dare maggior risalto a quanto sta accadendo in quell'area industriale. Oggi qui, in Senato, rinnovo la nostra disponibilità completa e totale a fare chiarezza definitiva su ambiguità, ombre e responsabilità sulla gestione degli accordi Golden Lady, collegati evidentemente, come si può capire anche dagli accadimenti di questi giorni, a responsabilità, disinteresse e leggerezze ministeriali. La chiusura dello stabilimento di Gissi ha prodotto il licenziamento di 382 lavoratori, in maggioranza donne, come conseguenza della delocalizzazione della produzione in Serbia, come già operato per la Omsa di Faenza (che peraltro è della stessa proprietà). Presso il Ministero dello sviluppo economico è stata concordata e condivisa unanimemente la proposta di nuova industrializzazione del sito di Gissi. La legge di stabilità del 2013 non ha previsto il finanziamento della formazione *on the job* che era alla base dell'accordo di riconversione raggiunto presso il Ministero. Per tale motivo lavoratrici e lavoratori sono quindi costretti ad un lunghissimo periodo di cassa integrazione. Le proposte, unitamente alla volontà di trovare soluzioni anche agli impegni dei diversi livelli istituzionali, funzionali e a rapido insediamento dei nuovi investitori, sono state sottoscritte anche dall'unità per la gestione delle vertenze del Ministero dello sviluppo economico, dai politici locali, da organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di categoria (CGL, CISL e UIL), oltre che dalle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali. sanno i lavoratori - è l'unica forza d'opposizione presente in Parlamento. Sarebbe un bene - da qui il mio invito - che tutti i parlamentari abruzzesi si unissero a noi del Movimento, quantomeno - come ho fatto con una interrogazione al Senato, la cui risposta peraltro attendo da tre mesi - nel richiedere al Ministero del lavoro di riconvocare le medesime parti firmatarie del verbale degli accordi sottoscritti, per ricomporre in maniera responsabile, definitiva, completa e certa il quadro degli impegni che risulta da più parti disatteso, anche in modo grave e unilaterale,